la posizione dell’Italia e di molti Paesi europei a proposito di un accostarsi della Turchia all’Unione Europea. Dunque, non eun episodio casuale avvenuto perche´ ad un certo punto a qualcuno andava di stabilire un rapporto di coproduzione cinematografica; evidentemente, c’e un incontro di attenzione e di reciproco interesse culturale da parte di coloro che si occupano di cultura in generale, e di cinema in particolare, nell’uno e nell’altro Paese.

di strutture, di organizzazione, di modo di intendere il valore culturale del cinema, di stabilire le rispettive responsabilita;

dell’Accordo. Vi sono numerose situazioni nelle quali si ricorda che si sta facendo insieme qualcosa che non puo che essere a beneficio della cultura

un ulteriore tassello dell’intensa relazione che lega l’Italia alla Turchia, in un’ottica che vede i due Paesi collaborare sempre piuattivamente, oltre che nel settore politico ed in quello economico, anche in quello socio-culturale. L’Italia e la Turchia rappresentano, del resto, due grandi aree di riferimento del Mediterraneo, depositarie di patrimoni culturali che hanno molti punti in contatto. L’Accordo di coproduzione cinematografica si inserisce, pertanto, in tale importante contesto bilaterale, come richiamava adesso anche il senatore Colombo, consentendoci di disporre di un quadro di riferimento anche normativo per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi in questo settore. L’avvio di una collaborazione nel settore sara sicuramente di grande rilievo per contribuire a quella migliore conoscenza reciproca, che siamo impegnati a promuovere, nelle sue varie forme e ai diversi livelli (Regioni, enti locali, associazioni), nella consapevolezza che essa costituisca strumento essenziale ad accompagnare il percorso di adesione della Turchia all’Unione Europea, tema – come e` noto – al centro del dibattito interno ai Paesi dell’Unione stessa.

in Commissione esteri – come ricordava poco fa il collega Pianetta – l’importanza di questo Accordo sulla coproduzione audiovisiva tra la Repubblica di Turchia e il nostro Paese.

E[]un Accordo che si colloca in un momento particolare. La Bulgaria e ormai entrata nella prospettiva di adesione all’Unione Europea, di cui ediventata Stato membro lo scorso gennaio. ovvio procedere, anche in questo caso, ad un aggiornamento degli Accordi precedenti, firmati nel 1963 e nel 1970. Questo Accordo e diretto ad ottimizzare le collaborazioni e le attivitadi scambio, gia avviate e regolamentate, e soprattutto a definire il complesso delle relazioni bilaterali, ai fini del rafforzamento dei rapporti di amicizia e del miglioramento della reciproca conoscenza. Nel merito, le due parti enunciano la volontadi perseguire forme di collaborazione, anche nell’ambito dei programmi promossi dall’Unione Europea, dall’UNESCO e dal Consiglio d’Europa, individuando i settori di comune interesse; tra questi si segnalano, in particolare, cultura, istruzione, scienza e tecnologia, ma anche temi piu specifici, quali la tutela dei diritti d’autore e la cooperazione in campo bibliotecario, librario e archivistico. Si prevede, inoltre – cosa molto significativa – la cooperazione tra le istituzioni culturali universitarie dei due Paesi e lo scambio di artisti, di esperti e di studiosi. Nell’ambito dell’Accordo, grande rilievo epoi assegnato all’esigenza di contrastare il traffico illecito di beni culturali, attraverso azioni di prevenzione e repressione, in conformita alla normativa nazionale e nel rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede internazionale. Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, composto da 4 articoli (che riguardano l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l’entrata in vigore), segnaliamo, in particolare, l’articolo 3,

Questo consentiradi favorire le attivita di scambio culturale – come abbiamo ricordato – e di assicurare il funzionamento della citata Commissione bilaterale proposta e la definizione dei programmi esecutivi. Proponiamo, pertanto, di approvare il provvedimento in esame.

stenografico 11 aprile 2007 aggiornato per le iniziative di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, nonche´ per lo sviluppo bilaterale degli scambi di tipo artistico, scolastico e di ricerca tra i due Paesi, come ha giaricordato poc’anzi il senatore Mantica. Lo scopo primario dell’Accordo e quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due Paesi attraverso lo scambio di esperienze e di dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo, al contempo, una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana in Bulgaria. Si tratta, in altri termini, di adeguare gli strumenti necessari per l’attuazione di una politica in campo culturale, scientifico e tecnologico verso un Paese con il quale da tempo l’Italia intrattiene rapporti privilegiati ed il cui recente ingresso nell’Unione Europea apre ulteriori ampie prospettive di collaborazione. La ratifica di tale nuovo strumento pattizio contribuiraalla realizzazione, nei rapporti con la Bulgaria, di un quadro normativo piu moderno, completo ed efficace, concorrendo cosıa rafforzare la gia eccellente cooperazione esistente tra i due Paesi.

luogo, perche´ la Bulgaria eentrata nell’Unione Europea e quindi questo Accordo ha la capacita e la possibilita` di rafforzare ulteriormente

lingua e di cultura italiana. Quindi, credo che questa sia un’opportunitache il nostro Paese ha a disposizione, per far sı che tutta la nostra capacita` di esprimere cultura, anche attraverso l’apprendimento della nostra lingua in terra bulgara, costituisca un elemento che rafforzi ulteriormente i rapporti e la coesione

Discussione delle mozioni nn. 51 della senatrice De Petris ed altri, 68 del senatore Polledri ed altri, 82 del senatore Marcora ed altri e 91 del senatore Scarpa Bonazza Buora ed altri, sull’industria agro-alimentare.